Onorevoli colleghi, si è conclusa da poco la Conferenza dei Capigruppo. Annuncio che la lettura e l'approvazione del calendario avverranno alle ore 17,30, salvo eventuali brevi differimenti in relazione all'andamento dei lavori.

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini

1, è volto a disciplinare il funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali, Il termine contenuto nella disposizione che consentiva al prefetto di designare i componenti aggiunti di quelle commissioni, in assenza dei componenti effettivi, fissato al 31 dicembre 2010, non è stato prorogato. L'esigenza di reintrodurre una disciplina compiuta al riguardo risiedeva dunque nella necessità di assicurare, già dal 16 aprile, in vista dei turni elettorali di primavera, la presenza dei componenti aggiuntivi delle commissioni, in assenza dei quali

L'introduzione di tale agevolazione colma una lacuna irragionevole nell'ordinamento, essendo già previste dalla normativa vigente agevolazioni per gli spostamenti marittimi e ferroviari. L'articolo 2 assicura la partecipazione al voto per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali. Tale norma consente a molti cittadini elettori di poter esercitare il diritto

ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, temporaneamente all'estero, ai professori e ai ricercatori universitari in servizio all'estero presso istituti di ricerca; Vengono dettagliatamente definite le condizioni per l'esercizio di tale diritto, con particolare riguardo all'onere di presentazione di un'apposita dichiarazione, da parte degli interessati, cui seguono adempimenti burocratici a carico delle amministrazioni di appartenenza dei votanti. Il comma 7 dell'articolo 2 estende a questo tipo di fattispecie, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sul voto degli italiani all'estero e del relativo regolamento di attuazione. Il comma 10 disciplina le modalità di scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero con quelle votate dagli elettori che risiedono all'estero stabilmente. L'articolo 3 stabilisce, infine, il termine di entrata in vigore del presente decreto-legge. La Commissione ha esaminato il decreto-legge nelle sedute del 13 e 20 aprile e del 3 maggio scorso. *(Brusìo).* PRESIDENTE. Scusate colleghi, per cortesia: non mi costringete a sospendere nuovamente la seduta. Io peraltro non ho grande propensione per la materia elettorale in questa giornata, signora Presidente, quindi lo faccio proprio per obbligo d'ufficio.

Pur condividendo la *ratio* delle proposte, ritengo di dover ribadire in questa sede l'invito al ritiro e a considerare le pur comprensibili esigenze in un'altra sede,

è comprensibile che l'attenzione di tutti noi sia ancora mentalmente assorbita dai risultati elettorali, però non possiamo trattare un provvedimento in materia di diritto di voto dei cittadini al *referendum* (a prescindere anche dai prossimi concreti quesiti che abbiamo di fronte a noi) come se fosse irrilevante o secondario, perché si tratta dell'esercizio del diritto di voto in una materia molto delicata, che dà un potere importante ai cittadini. Vorrei ricordare un passaggio di un discorso tenuto da Aldo Moro in Assemblea costituente il 16 ottobre del 1947 sul valore del *referendum*. Dice Aldo Moro, difendendo il testo: «Il presupposto dal quale partiamo nell'atto di stabilire, come abbiamo stabilito stamane, il *referendum* è questo: la possibilità di un disaccordo, fra la coscienza pubblica e le Camere che di essa dovrebbero tener conto nell'attività legislativa. Quindi, è inutile richiamarsi alle Camere, è inutile dire che esse intendono bene qual è il loro dovere di fronte ad una legge la quale non corrisponde alla coscienza pubblica. Ammettere il *referendum* significa ritenere appunto la possibilità di questo disaccordo, la possibilità di questa minore comprensione da parte delle

a una legge votata dal Parlamento. Per tale motivo ci rendiamo conto della situazione temporale in cui siamo e della difficoltà di introdurre emendamenti per questa concreta scadenza referendaria.

scusate se insisto, ed è veramente sgradevole costringermi ad essere così petulante. Credo, però, che il senatore Ceccanti, come prima il relatore, abbia diritto a svolgere le proprie argomentazioni La prima esigenza è quella dell'*election day*. Nel 2009 fu fatto l'abbinamento con il ballottaggio delle amministrative. Ora, prendiamo sul serio quanto affermiamo, di cui anche nelle scorse settimane abbiamo parlato, rispetto al debito pubblico. Non ha alcun senso rispetto al debito pubblico spendere anno dopo anno cifre intorno ai 300 milioni di euro per evitare l'abbinamento. Oltre tutto, negli altri Paesi europei, e anche negli Stati Uniti dove si pratica in maniera intensiva

Non c'è alcuna ragione per cui, prendendo sul serio il senso dell'articolo 75 della Costituzione, non si debba favorire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini. Se poi i cittadini anche in caso di *election day* non vogliono contribuire al *quorum*, possono sempre rifiutare la scheda e quindi decidere deliberatamente di non far scattare il *quorum*. Ma è importante non negare *a priori* questo diritto ai cittadini ed evitare che non sia preso sul serio quanto fecero i costituenti quando votarono l'articolo 75.

in effetti, dopo l'intervento del senatore Ceccanti, cade a proposito l'illustrazione del nostro ordine del giorno, il quale parte appunto con il primo articolo della Costituzione: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». La Costituzione ha previsto fin dall'inizio che il cittadino possa partecipare all'attività legislativa utilizzando due schede: con una scheda elegge i propri rappresentanti nel Parlamento e con l'altra, in caso, li corregge con il *referendum*, e in particolar modo con quello abrogativo. Bene, la legge applicativa del *referendum* è arrivata soltanto il 25 maggio 1970, quindi dopo oltre vent'anni dall'entrata in vigore della Costituzione. Tanto tempo è dovuto passare per avere una legge istitutiva. la convenzione antireferendaria in realtà vede tutta un'altra serie di applicazioni. Come radicali abbiamo scritto un testo che in vario modo abbiamo diffuso - lo abbiamo consegnato ai parlamentari, ma in ogni caso è rintracciabile sul sito Internet dei radicali - che si chiama

che dà un'interpretazione estensiva dei limiti per cui fare o non fare *referendum*. Ma soprattutto, il *referendum* si è visto svuotato nel momento in cui cittadini hanno votato per dei *referendum* e poi si sono viste leggi, approvate dal Parlamento, che andavano nella direzione esattamente opposta. Due casi per tutti: la responsabilità civile dei magistrati e il il finanziamento pubblico ai partiti. Inutile poi ricordare che dal 1990 non si raggiunge più un *quorum* nelle consultazioni referendarie, visto l'abbinamento tra i contrari a un *referendum* e chi, invece, per disaffezione, non partecipa più alle Il nostro ordine del giorno chiede tre impegni, che riassumo con tre *slogan*, praticamente, per restituire ai cittadini il compito di vigilare sul lavoro delle istituzioni, attraverso proprio la possibilità di emendare e di cancellare le decisioni del potere legislativo: l'abolizione del

dobbiamo convertire il decreto sulla scadenza referendaria. Lo faremo, ma questo è in contrasto logico-politico con l'operazione di dilazione del voto referendario che è stata messa in moto da qualche tempo. Noi obbediamo a un obbligo di legge nello stesso tempo, il Parlamento fa in modo di annichilire l'operazione sostanziale. La dilazione del voto referendario contiene in sé anche un elemento economicamente scandaloso, perché la maggioranza, che si fa forte della severità del Tesoro nel rispettare l'esigenza dei conti pubblici, accetta di condurre un'operazione per cui lo Stato spenderà circa 300 milioni in più, al solo scopo di tenere distinta la scadenza del voto referendario dal voto amministrativo. La modificazione del provvedimento riguardante il nucleare rappresenta un ulteriore motivo di scandalo. È giusto, legittimo che le Camere intervengano sulla materia in modo appropriato. Un *referendum* pone un problema, il Parlamento può ritenere di risolverlo in altro modo, e lo fa. Ma ciò che è stato iniziato su questo tema non è invece questa operazione, perché la modificazione del provvedimento su cui insiste il quesito referendario è una modificazione ipocrita, finge di modificare la norma mentre in realtà, per bocca del Capo del Governo, pubblicamente, si dice che, in realtà, è soltanto un mero rinvio della questione, per poterla affrontare con maggiore maturità tra un anno o due. Questo configura un tentativo surrettizio di impedire il pronunciamento del parere popolare su un tema di grande interesse, che viene in questa maniera, da una parte, dilazionato e reso più costoso e, dall'altra, reso sdrucciolevole per la dubbiosità della situazione in cui ci si viene a trovare. Si determina così un effetto, questo sì psicologicamente già accertato, che noi combattiamo ma che, invece, nella società, purtroppo, esiste. con la potenza adeguata dei mezzi di comunicazione si può far passare il principio che il quesito è stato comunque reso vano dall'opera della decisione del Governo e che, quindi, a questo punto, il *referendum* non ha più senso. il cinismo strumentale con cui è stato annunciato il rinvio del tema referendario ha la funzione la funzione di riuscire a determinare una sorta di tentativo per impedire il raggiungimento del *quorum*. Questo tentativo per impedire il raggiungimento del *quorum* è una ulteriore lesione alla possibilità del pronunciamento popolare sui quesiti referendari, come già la collega Poretti ha accennato nel suo intervento precedente. Inoltre, il tentativo di impedire il raggiungimento del *quorum* sul quesito referendario relativo al nucleare, trae con sé il tentativo di impedire lo stesso raggiungimento del *quorum* anche per il referendum sull'acqua e per quello sul legittimo impedimento, che rappresenta uno dei punti davvero dolenti degli interessi del Capo del Governo.

di discussione relativa alla partecipazione dei cittadini alle elezioni, quindi in una forma ambigua, mentre non può essere invece tenuto,

a proposito del *referendum* sul legittimo impedimento che, come sappiamo, serve a sottrarre il Presidente del Consiglio alle numerose azioni giudiziarie che egli si è meritato con la sua disinvoltura affaristica. poi qualche cosa che accentua la drammaticità della questione. La questione del nucleare è resa ora ancora più centrale dal fatto che, per iniziativa stessa

grande partecipazione al voto e rifiuto totale della prospettiva del nucleare. Si tratta di un tema sul quale la maggioranza dovrebbe interrogarsi senza alcuna sollecitazione, perché è un problema che la pone di fronte ad una contraddizione assolutamente trasparente: in effetti, mentre il Governo vuole a tutti costi il nucleare e vuole in qualche maniera imporlo alle Regioni, una Regione

che aveva costituito il paradigma che rendeva difficilissimo sostenere le ragioni di nuove azioni sul piano nucleare, è scomparsa dall'orizzonte della comunicazione pubblica,

C'è il silenzio colpevole della RAI che, vincolata da delibere della Commissione di vigilanza, dalla legge, dal sentire comune dovrebbe offrire ai cittadini una informazione accurata, completa, scientificamente attendibile, significativa nel proporre le varie possibilità di opzioni, ha invece consegnato pochissimi, asfittici elementi di informazione e di comunicazione su questo piano in alcune reti e non in tutte, ed in orari impossibili. Ciò significa che la questione dei *referendum* non solo è attaccata sul piano del tentativo di dilazione colposo e costoso e truccando le modificazioni dei provvedimenti su cui insiste il quesito referendario, ma è anche attaccata con un silenzio plumbeo, volontario, che si attiva ovviamente e per forza di cose sulla base del potere di influenza che il Governo estende sulle reti pubbliche a causa della propria presenza di maggioranza. È una situazione pericolosa perché la democrazia è fatta di consapevolezza e di informazione. Noi assistiamo ad un momento importante della decisione pubblica su un argomento significativo e non c'è consapevolezza e informazione, ma annebbiamento e tentativo di rendere opaco tutto il meccanismo della conoscenza su questo piano. Credo che questo debba essere considerato con attenzione da chiunque abbia a cuore la possibilità dei cittadini di esprimersi nella completezza dei propri mezzi intellettuali.

senatore Pardi ha parlato di dilazione e di opacità. Io direi che più che di dilazione qui si deve parlare di vera e propria cancellazione, e più che di opacità parlerei di oscurità. Ci sono state ripetute sedute della Commissione bicamerale di vigilanza - che dovrebbe, oltre che aprire un occhio su come viene gestito il servizio radiotelevisivo pubblico, anche indirizzarne addirittura la programmazione - che non sono riuscite a a fare adottare in tempo utile il regolamento: utile non perché lo dicono coloro i quali sostengono il sì o la necessità di andare a votare sui *referendum*, ma perché la legge prevede che, entro il 4 aprile di quest'anno, il regolamento avrebbe dovuto consentire l'informazione istituzionale nonché l'apertura dei contraddittori.

nelle televisioni e nei telegiornali, con il risultato che in 10 si dividono tutto lo *share*, dalla mattina alla sera. L'ordine del giorno G.100 denuncia proprio il fatto che il regolamento è stato approvato il 5 maggio scorso e che avrebbe dovuto entrare in vigore ieri, il 16 maggio, cioè a meno di di un mese dallo svolgimento dei *referendum*. Questo va contro tutti i diritti costituzionalmente garantiti, non soltanto di libertà d'informazione, ma anche di fare informazione nel merito, oltre che nel merito, su questioni che, com'è stato ricordato in esordio dal senatore Ceccanti, costituiscono l'unica arma democratica e di partecipazione diretta consegnata ai cittadini dai Costituenti, cioè la scheda referendaria. Questo lo si afferma non perché, ripeto, si vogliono votare quattro «sì» ai quattro *referendum* (e questo lo dice un radicale che, proprio nella prima campagna referendaria del 1974, sostenne il *referendum* per andare a votare «no»: furono i «no» a vincere in quella tornata referendaria per confermare la legge che legalizzava il divorzio in un Paese in cui si riteneva che gli italiani non fossero ancora pronti ad affrontare quelle questioni). Le questioni che ci aspettano da qui a tre settimane sono altrettanto complesse e occorre che - questo è quello che chiediamo al Governo - si recuperino tutti gli spazi, non solo all'interno delle soporifere tribune referendarie, ma anche nelle trasmissioni di massima informazione, nelle fasce di massimo ascolto e anche nelle presunte trasmissioni di intrattenimento e approfondimento che, ancora una volta, faranno di tutto per espellere dal dibattito i *referendum*.

programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti, esprime, altresì, parere non ostativo ad eccezione che sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.0.1, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dichiaro improponibile l'emendamento 1.0.100 in quanto estraneo all'oggetto del decreto‑legge in esame che reca unicamente disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni di viaggio, nonché in materia di voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali in occasione delle prossime consultazioni referendarie. Passiamo all'esame

Ricordo infatti che la legge n. 352 del 1970 inibisce esclusivamente la contemporaneità di svolgimento dei *referendum* con le elezioni politiche e che tutti noi ci siamo impegnati in queste ultime settimane nell'ambito della discussione del Piano nazionale di riforma a fare delle scelte tali da non incrementare il debito pubblico.

il nostro emendamento, di cui sono prima firmataria, tendeva a operare un intervento sulle recenti elezioni amministrative. In che senso?

Grazie Veniamo adesso da una tornata amministrativa e da questo voto a Milano (che ci ha dato anche qualche soddisfazione, se mi permettete di dirlo in questa sede):

andare a una consultazione popolare. Ciò è avvenuto per una norma di legge (purtroppo non ero tra i legislatori, quindi non so ricostruire a quale *ratio* corrispondesse)

in questo clima in cui gli elettori ci guardano aspettando segnali di contenimento della stessa (dove

per facilitare l'espressione di voto popolare sui quesiti referendari. Non ripeto le parole del senatore Ceccanti sull'istituto così come introdotto nella Costituzione e

Presidente, i risultati elettorali si prestano a qualche discussione, lo capisco.

di introdurre una norma che abolisse tale divieto, permettendo lo svolgimento e suggerendo di andare al ballottaggio esattamente come viene fatto per i quesiti referendari di interesse nazionale: ciò, sia per ragioni di spesa, sia per favorire al massimo la partecipazione dei cittadini, e non - invece - ostacolarla. Se mi permette, signora Presidente, vorrei svolgere ancora una riflessione. Non si è voluto tenere conto di questo nostro emendamento quando è stato presentato in tempo utile per poter incidere già sulle amministrative. Forse qualcuno pensava che non si sarebbe mai andati al ballottaggio e che, quindi, sarebbe stato superfluo.

che ogni volta ricordano a tutti il ruolo del Parlamento, richiamando la maggioranza e il Governo a dare piena dignità e a facilitare in tutti i modi l'espressione referendaria. Noi siamo assolutamente convinti che un'istituzione come il Parlamento solo da guadagnare in credibilità rendendo i suoi lavori più snelli e più basati sulle funzioni legislative essenziali e ricostruendo con i cittadini attraverso queste forme di partecipazione. Noi abbiamo presentato un disegno di legge - anche questo depositato per tempo, tre anni fa, all'inizio della legislatura - per rendere più snello, ma anche

con intelligenza, per rendere più credibile il ruolo del Parlamento, che non ha paura dei *referendum*, ma anzi si affida su molte materie con fiducia ai cittadini.

stesse zone in cui si svolgono le missioni internazionali alle quali partecipa l'Italia equiparandolo al personale militare, dal momento che le missioni internazionali coinvolgono a vario titolo persone che svolgono un lavoro di importanza equivalente. A fianco

G2.0.1 fa riferimento agli studenti universitari fuori sede, i quali già in minima parte oggi votano nei luoghi in cui studiano

Signora Presidente, solleverò l'Aula dall'imbarazzo di starmi ad ascoltare con una dichiarazione di voto molto breve. Del resto, ho espresso le mie ragioni poco fa nell'intervento Il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà favorevolmente alla conversione in legge del decreto-legge, mantenendo intatte tutte le sue riserve di ordine logico-politico a proposito del tentativo riuscito, ahimè, di dilazione del voto referendario, a proposito dello scandaloso aumento dei costi che questa dilazione ha comportato, a proposito anche della modificazione ipocrita del provvedimento sul nucleare creata *ad hoc* per suggerire all'opinione pubblica l'inutilità del quesito referendario sul nucleare.

in un certo senso, nella prassi politica determinata dal Governo e dalla maggioranza nel mese precedente, delle ragioni profondamente contraddittorie. Noi stiamo lavorando per realizzare un *referendum* che la maggioranza si è impegnata attivamente a svuotare il più possibile, allontanando i cittadini dalla consapevolezza e dalla conoscenza e rendendo democraticamente difficile la realizzazione di un diritto democratico.

ma desidero anche sottolineare l'errore che è stato fatto nel non accorpare in un solo giorno il *referendum* e le elezioni amministrative. Questo avrebbe consentito di risparmiare almeno 300 milioni di euro e Dio solo sa quanto ci sia la necessità di contenere le spese. Pertanto, voglio sottolineare che l'Unione di Centro ha più volte

Resta il problema di quello che manca, ossia l'*election day*. Si sperperano 300 milioni di euro in un periodo in cui le nostre finanze pubbliche non se lo potrebbero permettere e non si è voluto neanche accettare quell'ordine del giorno che era importante per le consultazioni future. Speriamo che anche le consultazioni elettorali di questi giorni servano a capire che bisognerebbe sempre scegliere l'interesse del Paese, e 300 milioni sono un interesse molto materiale del Paese, che avrebbe meritato di essere preso in considerazione. Signora Presidente, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà sul provvedimento, voglio sottolineare l'importanza dello stesso, che consente agli agenti, ai funzionari in servizio all'estero e ai militari impegnati nelle missioni internazionali

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo riunitasi oggi pomeriggio ha approvato, a maggioranza, modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 26 maggio. Fermo restando l'esame dei decreti-legge già presenti in calendario, per i quali si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi, nel corso della settimana corrente saranno discusse la relazione sull'attività svolta dalla Commissione straordinaria per il controllo dei prezzi negli anni 2009 e 2010 e la risoluzione sull'atto comunitario concernente «Partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale». La prossima settimana il calendario prevede l'eventuale seguito dei decreti-legge non conclusi, la discussione dei la discussione dei disegni di legge in materia di rappresentanza locale degli italiani residenti all'estero, già rinviati in Commissione, il seguito della mozione Micheloni sulla razionalizzazione della rete diplomatico-consolare italiana, l'esame di ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione esteri e l'eventuale seguito di argomenti non conclusi. In relazione alle elezioni amministrative, la seduta pomeridiana di mercoledì 25 maggio avrà termine alle ore 19, ove concluso 1'esame dei decreti-legge in calendario. Il sindacato ispettivo è anticipato alla seduta antimeridiana di giovedì 26. Il calendario sarà inoltre integrato con la deliberazione dell'Assemblea sulla costituzione in giudizio per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Milano, con riferimento a una vicenda processuale riguardante l'ex senatore Iannuzzi. In relazione ai tempi di scadenza, la deliberazione avrà luogo prima del 25 maggio. La Conferenza dei Capigruppo ha infine preso atto delle determinazioni assunte dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relativamente alla vicenda processuale

questione più volte sollecitata che ad oggi non ha ancora trovato soluzione. Abbiamo dichiarato ripetutamente del Partito Democratico non avrebbe più votato a favore di calendari d'Aula nei quali non fosse stata inserita la discussione sul provvedimento anticorruzione.

difficoltà particolarmente pesante per i Gruppi di opposizione, che si trovano spesso nella impossibilità di chiedere la calendarizzazione di propri provvedimenti, fermi in Commissione da tempo immemorabile

prima, anticipata dal collega Zanda, riguarda la mancata calendarizzazione dei disegni di legge in materia di anticorruzione. Credo sia obiettivamente sconveniente - non voglio usare termini particolarmente forti - che la maggioranza si trinceri dietro il parere della Commissione bilancio.

candidati ed esponenti politici di diverso colore sono stati trovati con le mani nel sacco. Pertanto, l'idea di dare un segnale reale ed efficace inasprendo una serie di sanzioni sul fronte dell'anticorruzione sarebbe una una cosa di buon senso. Mi sembra però che il buon senso non aleggi dalle parti della maggioranza. La seconda ragione per la quale non abbiamo votato il calendario e continueremo a non votarlo riguarda l'assenza e il rifiuto del Governo e del ministro Maroni a rendere in Aula, su nostra richiesta, un'informativa, in occasione dell'esame del decreto-legge nostra richiesta, un'informativa, in occasione dell'esame del decreto-legge che riguarda la concessione *una tantum* di provvidenze e benefici in favore del personale del comparto sicurezza,

anche alle improvvide dichiarazioni del Ministro stesso in ordine alla sentenza della Corte costituzionale e alla decisione della Corte di giustizia europea in materia di ronde e di reato di immigrazione clandestina, ed anche per avere l'occasione per avere alcuni dati inerenti i procedimenti penali in corso per immigrazione clandestina, il numero delle espulsioni con accompagnamento alla frontiera effettivamente realizzate da tre anni a questa parte (grazie ai famosissimi pacchetti sicurezza della maggioranza), con riferimento al funzionamento delle norme, sempre contenute nel pacchetto sicurezza, che riguardano l'immediata espellibilità degli extracomunitari che siano ospiti ospiti delle nostre patrie galere e che siano stati condannati ad una pena superiore a due anni di reclusione. Per capire, cioè, se tutto quello che è stato fatto su questa materia è una "bufala" oppure se, dopo tre anni, ha trovato pratica attuazione.

di questa materia, cioè di sicurezza, se ne debba discutere in Aula, perché trattasi di materia d'interesse generale, credo che rifiutarsi di venire a rendere questa informativa sia un'ammissione di questo Governo circa il fatto che non è nelle condizioni di governare in termini di efficienza né il personale delle forze di polizia, La terza ragione per la quale noi non abbiamo votato il calendario è perché siamo contrari al ritorno in Aula - quindi all'esame e all'approvazione - del provvedimento che riguarda la disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero, perché riteniamo che sia un provvedimento gravissimo, sbagliato, che viola i principi di democrazia e di rappresentanza dei nostri connazionali residenti all'estero attribuendo un potere discrezionale al Governo nella selezione dei rappresentanti degli italiani all'estero. Queste sono le ragioni per le quali abbiamo votato contro il calendario e - lo dico

e ve ne spiego la ragione. Celebriamo in questi giorni il primo anniversario del Consiglio dei ministri straordinario in cui venne presentato il disegno di legge del Governo di anticorruzione. Fu un fatto eccezionale, perché convocato il Consiglio dei ministri di lunedì, casualmente in coincidenza con la data di un processo, perché era importante intervenire sulla materia della corruzione. É passato un anno; poi finalmente

del prodotto del Governo, abbiamo rinunciato alla discussione generale per spostare tutto in fase di esame degli emendamenti. Sennonché la maggioranza fa la pratica ostruzionistica al Governo: mentre noi cerchiamo di dare una mano al Governo, la maggioranza rallenta il lavoro. Nel mese di ottobre, esattamente il giorno 6 ottobre del 2010, gli emendamenti sono stati messi a disposizione della Commissione bilancio. Sono passati sette mesi sette mesi e mezzo, e ancora non si vede l'esito. É chiaro che questo è un atteggiamento ostruzionistico:

Ma questo fa il paio, signor Presidente e onorevoli colleghi, con il disegno di legge, presentato nel novembre 2008, di ratifica della Convenzione di Strasburgo del 1999

Sono mesi, signor Presidente, che il Governo chiede il rinvio perché deve fornire il parere su un unico ordine del giorno presentato in Commissione. Se questo non è ostruzionismo della maggioranza contro il Governo e del Governo contro se stesso, che cosa è? Perché sulla corruzione vengono posti tutti questi freni? freni? Per quale motivo non si riesce a portare in Aula un qualcosa che si era detto essere essenziale, anche alla luce delle denunce provenienti dalla Corte dei conti sul disastro che induce la corruzione sul nostro sistema economico? Insomma, vogliamo affrontare questa disciplina, oppure dobbiamo occuparci della prescrizione breve? È questo il problema. Noi vogliamo affrontare i provvedimenti anche proposti dal Governo su temi importanti che condividiamo, ma non possiamo subire una pratica ostruzionistica che non fa bene al Paese e non è nell'interesse dei cittadini.

per inserirvi l'informativa del Ministro dell'interno su questioni di sua competenza sia per espungere dal calendario il disegno di legge sulla rappresentanza degli italiani all'estero.

e ad espungere dal calendario il disegno di legge sulla rappresentanza degli italiani all'estero.

Passoni, Ghedini, Adamo, oltre che della sottoscritta. Con questa interrogazione intendiamo riportare all'attenzione dell'Aula e del Governo il tema della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari

Gli ospedali psichiatrici giudiziari avrebbero dovuto essere già tutti chiusi - le norme lo prevedono - fin dall'aprile del 2008. Invece, non soltanto in questi manicomi criminali - così si chiamavano una volta - ci sono 1.300 internati,

tragedia di sofferenza, di privazione, di negazione dei diritti umani e dei diritti individuali tutelati dalla nostra Costituzione. Non esiste nessun motivo per gli ospedali psichiatrici giudiziari debbano ancora rimanere aperti. Non ci debbono essere più dilazioni e per questo noi chiediamo che il Governo si attivi al più presto, in particolare che nomini commissari *ad acta* per definire tempi certi per la chiusura degli OPG. La preghiamo dunque, signora Presidente, di sollecitare il Governo affinché risponda

che dal 1996 impone dei tassi-soglia per tipologia di prestiti, oltre i quali un prestito diventa usurario. Questa legge prevedeva che, usura, ai tassi registrati nel trimestre precedente fosse aggiunta una percentuale del 50

il tasso di riferimento della Banca centrale europea. Ora - e concludo, signora Presidente - cosa è successo? Il Ministro dell'economia, nella norma considerata sviluppo - probabilmente si riferiva allo sviluppo dei banchieri con i quali va a braccetto - ha modificato questi tassi-soglia, quasi a fare la politica monetaria che spetta alla Banca centrale europea, per cui i mutui a tasso variabile subiranno incrementi dell'80 i mutui a tasso fisso subiranno incrementi del 60 per cento. Questo lo chiamano sviluppo: probabilmente, si degli interessi dei banchieri, non certo quelli delle famiglie che fanno fatica a pagare le rate dei mutui. Allora - la ringrazio e concludo, signora Presidente che si risponda a queste interrogazioni (sono tante) che continuerò a sollecitare, e che questo Governo la smetta di andare sottobraccio ai banchieri. Ricordo che il ministro Tremonti, in una audizione alla Commissione finanze, affermò che i banchieri che sbagliano o vanno a casa o vanno in galera; invece, sono tutti a piede libero. Il ministro Tremonti ricorda quella storia dei ladri di Pisa: fanno finta di litigare di giorno